Comunico che in data 11 gennaio 2019 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia* «Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi» (1002).

La Conferenza dei Capigruppo ha adottato modifiche al calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 7 febbraio. In relazione ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 8a, la discussione del decreto-legge semplificazioni inizierà martedì 22 gennaio, con seduta dalle ore 9,30 alle ore 22. è stata rimodulata la ripartizione dei tempi di discussione tra i Gruppi. La settimana corrente sarà pertanto dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni. Resta confermato per giovedì confermato per giovedì 17 alle ore 15 il *question time*, con la presenza dei ministri Salvini, Bussetti e Fontana. Mercoledì 23 gennaio, alle ore 16, sarà discussa la relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

delle Commissioni. Nella settimana dal 5 al 7 febbraio saranno discussi il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge sull'applicabilità delle leggi elettorali, sulla videosorveglianza e la ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di confermare nella sessione annuale del 2019 la delegazione dei senatori attualmente in carica presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Mercoledì 23 gennaio, alle ore 8,30, saranno convocate, per la loro costituzione, le Commissioni bicamerali semplificazione e questioni regionali, mentre giovedì 24 gennaio, alle ore 8,30, saranno convocate le Commissioni vigilanza anagrafe tributaria e controllo enti gestori. Sempre nella giornata di giovedì 24 gennaio, alle ore 8,30, sarà convocato il Consiglio di garanzia.

Governo sta infliggendo all'Italia, sulle conseguenze per la nostra economia, sulla nostra crescita o meglio - come abbiamo capito con molta chiarezza recentemente - sulla nostra di questo dibattito esiste la questione importante, anzi importantissima, relativa all'intervento sulla TAV, una questione che conosciamo molto bene da tanti anni, su cui tanti Governi e tante maggioranze si sono espressi. Nel

Visto che la maggioranza ha piacere, ha gusto, prova divertimento nel continuare a prendere in giro gli italiani sui giornali, con i *media,* sui *social network* prendendo le posizioni più diverse e cercando di creare una confusione, o piuttosto una cortina di fumo per cui mai si capisce effettivamente cosa pensi, noi abbiamo chiesto un atto molto semplice di trasparenza, di chiarezza nei confronti dell'Italia e di quello che noi ci aspettiamo per l'Italia dal futuro. Il Governo deve avere il coraggio di esprimere le proprie decisioni e le forze politiche che lo sostengono devono avere il coraggio di venire nella sede propria, il Parlamento italiano, e dirci cosa pensano sul futuro della TAV. Il Partito Democratico ha chiarezza rispetto a questo, ha presentato la mozione n. 65, che chiediamo di calendarizzare in questa settimana,

nascondersi dietro il fumo di strane Commissioni, fatte *ad hoc* per cosa? Per dare un giudizio di merito? No, per guadagnare, anzi, per far perdere mesi e mesi agli italiani, all'Italia e alla nostra economia,

proposto dal Governo, anzi disposto e poi riorganizzato da un Governo che non è in grado di darsi un calendario dei lavori che possa rispettare. Gruppo FI-BP)*. Vogliamo sottolinearlo, colleghi, perché non è solo forma: sappiamo che in politica, soprattutto in queste Aule parlamentari, la forma è sostanza. Quello che abbiamo detto e diciamo come Gruppo parlamentare e che vogliamo ribadire anche all'esterno di quest'Aula, è che non può essere scaricata sulla minoranza la responsabilità di provvedimenti che sono sempre in ritardo e vengono

L'apposizione della fiducia rappresenta una difficoltà del Governo di rimanere associato con se stesso. Questo è il motivo, signor Presidente e colleghi, per cui noi abbiamo votato contro questo calendario del lavori. Un altro motivo? Anche noi abbiamo presentato delle mozioni. Anche noi abbiamo presentato una mozione a cui teniamo massimamente: la mozione per favorire la prosecuzione dei lavori della TAV, dell'Alta velocità Torino-Lione, a cui non solo noi, ma tante tante categorie produttive da non poter essere ignorate ricollegano il futuro, il benessere e il prosieguo dello sviluppo economico del Paese. Ci sono stati degli impegni, anche istituzionali, forti delle Assemblee parlamentari. Noi abbiamo presentato una nostra autonoma mozione, come Forza Italia, perché rivendichiamo l'originalità e l'univocità della posizione sulla TAV, sempre

siamo stati sempre a favore dell'Alta velocità. Noi siamo quelli della legge sulle grandi opere. Noi siamo quelli dell'Alta velocità realizzata, non raccontata. Noi siamo quelli che non hanno mai cambiato idea a seconda delle zone in cui andavano a raccontare dell'Alta velocità. Noi abbiamo detto sì a Torino, come in Val di Susa, a differenza di alcuni Presidenti di Regione piemontesi che invece cambiavano idea a seconda del territorio che si trovavano ad arringare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ed è questo il motivo per cui noi chiediamo e rivendichiamo la calendarizzazione di una mozione autonoma di Forza Italia, che ha sempre detto sì e creduto fortemente nell'Alta velocità. A questo proposito, colleghi - e con questo concludo, signor Presidente, perché rappresenta un'ulteriore richiesta da parte di Forza Italia - vorremmo sollecitare la calendarizzazione di una mozione che tenga conto di parole che non possono essere ignorate: le parole che il Presidente della Repubblica ha pronunciato - non farò il suo nome, rivendicando il suo ruolo di terzo garante della Costituzione, ha acceso un riflettore sulla difficoltà di avallare procedure come quelle che ha subito

con una serie di considerazioni a dir poco suggestive per il futuro, ossia la possibilità per ciascun parlamentare di fare ricorso direttamente alla Corte costituzionale e soprattutto

ufficialmente, a nome del mio Gruppo, la calendarizzazione di una mozione che tenga conto di questi elementi, oltre che di altre due mozioni, da tempo in attesa di essere calendarizzate, sull'autismo e su altre disabilità e sui Comites, ossia cittadini italiani eletti all'estero che da sempre si sono costituiti in organismo organizzato, anche nelle legislature precedenti.

dal Presidente del Gruppo Partito Democratico ed ora dalla Presidente del Gruppo Forza Italia, forte di un convincimento che deriva da un'esperienza che nelle Aule parlamentari non è mai venuta meno, salvo che nell'ultima discussione sulla legge di bilancio. In genere, in sede di discussione sulla manovra finanziaria, si allega anche un piano delle opere infrastrutturali di cui il Paese abbisogna. Noi abbiamo vissuto un momento particolarmente negativo nell'ultima discussione, quando quel piano non è stato allegato. E oggi non sappiamo, salvo avere la certezza che 24 miliardi di lavori siano stati bloccati dall'attuale Governo, quali siano le priorità del Governo Salvini-Di Maio nel dare esecuzione ad opere di cui il Paese ha bisogno; 24 miliardi di lavori bloccati e la TAV è tra questi. È questa la ragione per la quale una discussione rapida, tanto meglio nel corso di questa settimana, del tema che riguarda la TAV e le grandi opere pubbliche a oggi bloccate non possa

in quest'Aula votò a favore dell'accordo internazionale italo-francese che metteva la parola «fine», accanto ad una serie altra di fatti e di provvedimenti, al tema dell'Alta velocità Torino-Lione. Oggi viene rimesso in discussione: è giusto che l'Assemblea riesamini la questione e fermi il punto, perché l'opera è decisamente significativa per il nostro Paese.

di non trattare l'argomento, anzi noi non abbiamo mai nascosto che la Lega è a favore dell'Alta velocità, ma giustamente abbiamo sottoscritto un contratto di Governo con i nostri *partner*, nel quale si prevede una revisione dell'opera alla luce di un'analisi un'analisi costi-benefici, quindi con perfetta coerenza noi ci comportiamo in questo modo. Quando arriverà l'analisi costi-benefici, saremo pronti e arriveremo molto probabilmente con una mozione di maggioranza ovviamente, sarà figlia di un accordo e di un compromesso su questo tema importante da parte della formazione di Governo. Signor Presidente, io penso invece che l'azione che questo Governo sta facendo da qualche mese, da quando governa il Paese, sia molto chiara rispetto agli investimenti. Porto ad esempio la norma cosiddetta spagnola, quella che ha dato 400 milioni di euro ai piccoli Comuni, che fanno quelle opere utili per il nostro tessuto tessuto e per i nostri cittadini, quei piccoli Comuni che non avevano soldi per fare assolutamente niente e che grazie a questo Governo e a questa maggioranza oggi, in poco tempo, potranno mettere in campo degli interventi infrastrutturali molto utili per i cittadini. invece molto perplessi sulla questione delle grandi opere quando sono grandi opere inutili, non quando sono grandi opere utili ed è questo che abbiamo sottolineato. dal punto di vista della maggioranza, come sottolineato più volte in questi giorni, il contratto di Governo prevede una cosa molto semplice: non aspettare un documento inutile da qualche commissione inutile, come qualcuno ha detto testé, ma attendere una commissione seria, che è stata fatta dal Ministero, per capire l'analisi costi-benefici di quell'opera e sulla base di quel dato portare anche in quest'Aula la discussione sulla realizzazione dell'opera. Rispetto ad altri temi che sono stati toccati, credo che quello che stiamo cercando di fare sul decreto semplificazioni sia un'altra azione utile per un Paese che, se ha bisogno di così tante semplificazioni, è perché in questi anni lo avete complicato un po' troppo. Il fatto che diventi un documento corposo è legato a questo, perché chi ha governato prima di noi evidentemente ha complicato la vita dei cittadini. Cerchiamo di semplificargliela e lo faremo seguendo una procedura ordinaria, lavorando nelle Commissioni e giungendo in quest'Aula la prossima settimana con il decreto semplificazione.

oggetto specifico, sul quale vorremmo essere chiari, se non lo fossimo già stati, a nostro avviso, abbondantemente. Mi riferisco alla questione TAV, che è stata citata da alcuni colleghi che sono intervenuti. Intanto vorrei ricordare a questa Assemblea, ma anche fuori, che la nostra presidente Giorgia Meloni chiese al sindaco di Torino, in tempi si direbbe non sospetti, un *referendum* per far scegliere ai cittadini cosa fare rispetto alle

ma rafforza una posizione come quella di Fratelli d'Italia, che è molto chiara: noi eravamo anche sabato scorso in piazza a Torino, per dire che siamo favorevoli alle grandi opere, siamo favorevoli alle infrastrutture, siamo favorevoli alla TAV,

dice di voler fare un non ben definito *referendum* e l'altra parte del Governo risponde che il *referendum* non conta ma conta il contratto e quello che c'è scritto. questo è un problema vostro, brutalmente: sono affari vostri. Noi, invece, pensiamo che quest'Aula debba esprimersi sul tema, debba entrare nel merito e debba discutere, perché siamo stanchi di votare votare ad occhi chiusi provvedimenti che arrivano in ritardo e, almeno su questo, vorremmo anticipare le conclusioni di una commissione di valutazione costi-benefici nella convinzione che sia la politica che deve valutare i costi e i benefici. Comunque, la commissione farà il suo lavoro ma quest'Assemblea deve discutere e confrontarsi e Fratelli d'Italia presenterà una sua mozione sul tema a favore della TAV e a favore delle grandi opere.

la mozione con cui il Partito Democratico chiede al Governo parole chiare sul destino del progetto per la realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione è persino più eloquente di un voto. Ci dice che la contrarietà all'opera è una posizione che la Lega non ha scartato o che non ha la forza o il coraggio di scartare perché mancano la forza e il coraggio di affrancarsi dalle contraddizioni con cui paga quotidianamente il suo ruolo di Governo. Il patto scellerato con l'alleato a 5 Stelle vale più dell'interesse generale, tanto che si sceglie di non scegliere e di mortificare le migliaia di persone che in un moto autenticamente referendario, esplicito ed ed inequivocabile per ben due volte in pochi mesi sono scese in piazza a Torino a invocare una decisione. C'era anche la Lega in quella piazza, c'era anche la Lega. Una piazza tradita in soli tre giorni nel nome di un potere che si dimostra cinico al punto da silenziare il pronunciamento di quest'Aula. Sia chiaro: costringere il Senato al silenzio con una furberia procedurale non è solamente fumo negli occhi di chi è andato in piazza, ma è mettere il bavaglio alla democrazia. c'è una contraddizione tra lei e il ministro Toninelli: mentre il ministro Toninelli ci chiede di aspettare ancora qualche settimana affinchè il Governo possa esprimere un giudizio sull'analisi costi-benefici, lei, in contraddizione anche con quello che ha detto oggi, cosa dichiara ai giornali? «Un sì alla Torino-Lione ci metterebbe in difficoltà perché la base», del vostro MoVimento, «non capirebbe. Ci sarebbe un problema di tenuta interna E di motivi nell'analisi costi-benefici non mi sembra che ce ne siano». Quindi siete arrivati a una conclusione:

potuto approfittarne in quest'Aula per spiegare agli italiani che l'Alta Velocità Torino-Lione non costa 20 miliardi. Avete un Ministro dell'economia che può spiegarvi che è una frottola raccontare agli italiani che stiamo spendendo 20 miliardi per la Torino-Lione: non è così. E una analisi costi-benefici, così come il piano industriale di un'azienda, si fa prima

il Gruppo Forza Italia naturalmente voterà a favore della proposta avanzata dalla sua Presidente, la senatrice Bernini, di calendarizzare nel breve termine le mozioni sulla linea ferroviaria ad alta velocità,

applica l'iperpoliticizzazione a qualunque tema: indipendentemente dalle posizioni, bisogna rinviare la decisione per evitare squilibri politici nella maggioranza.

siamo felici - vediamo la conferma che la commissione costi-benefici serve a dare un beneficio politico: ha sicuramente un costo per gli italiani, perché vuol dire perdere mesi perdere mesi di competitività e di lavoro effettivo (ci sono persone che prima lavoravano e che oggi non lavorano perché i cantieri sono stati fermati), ma i benefici sono unicamente di carattere politico per la maggioranza, la quale così si leva dall'imbarazzo di dire sì o no a una cosa che, comunque la si veda, è estremamente importante per l'Italia. Tant'è vero che chi si è schierato da una parte o dall'altra - ma direi soprattutto chi si è schierato dall'altra

possiamo ribadire che lo studio dei costi e dei benefici si fa prima di iniziare un'opera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Non si inizia l'opera, si arriva a un punto in cui ci sono già chilometri di galleria, anche definitiva, già costruita, nonostante qualche esponente del Governo

fortunatamente metaforica - bomba sotto quest'opera. Si tratta di un'opera che porterà occupazione nella costruzione, ma soprattutto - quello che più conta - dopo. Senza quest'opera il nostro Paese sarà tagliato fuori dalle grandi comunicazioni internazionali, dalla grande comunicazione dall'Ovest all'Est dell'Europa

con la valutazione più bassa. Stiamo parlando della nomina del direttore generale di un grande ospedale. Inoltre il contratto è stato sottoscritto in tutta fretta, con una delibera di designazione ancora non pubblicata, né nel bollettino ufficiale e neanche sul sito *on line* della Regione. Tale emergenza è tra l'altro immotivata, perché ci sono i commissari in carica e sono arrivate ben due diffide alla stipula. Tale fretta, quindi, sembra mirata solo a disarmare il ricorrente al TAR, per non permettere l'ottenimento della sospensione urgente delle procedure di assunzione. Ancora più grave è che

la Giunta, scaduta da tempo, che fa nomine dell'ultimo minuto e la facente funzione che trattiene la poltrona e rimanda le elezioni a maggio. Voglio però ricordare che il MoVimento 5 Stelle ha presentato ricorso al TAR,

periodo di proroga forzata del mandato, siano solo espressione della necessità di riempire gli organigrammi e, anzi, di occupare in fretta le ultime poltrone. È una vergogna! Siamo di fronte quindi ad una nomina politica in danno al merito? Siamo addirittura contro l'interesse della salute pubblica?

in essere ogni iniziativa che possa fare luce su tali eventi e monitorare continuamente l'evoluzione della gestione sanitaria lucana, che è e deve rimanere una sanità di eccellenza per la collettività lucana e non solo. Se posso aggiungere, ogni ogni azione delle istituzioni pubbliche fatta non nell'assoluto rispetto del diritto della salute del cittadino e in danno del merito e dell'efficienza deve essere sempre verificata, contrastata e vanificata.

combatte per vedere riconosciuti dei diritti. Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione e il concorso deve essere rifatto, perché non vi erano regole. Nel 2018 il Consiglio di Stato, nella medesima università, annulla un concorso in chirurgia generale. Nel 2018 il Consiglio di Stato annulla un concorso in diritto amministrativo. Nel 2018 il TAR annulla un concorso in urologia nella stessa università; e altri ricorsi sono pendenti. Non solo. L'attuale rettore è imputato per tentata concussione e istigazione alla corruzione. L'ex rettore, insieme all'attuale docente di diritto commerciale, sono indagati per circonvenzione di incapace, per aver convinto una ricca vedova a firmare atti che hanno concorso a privarla del controllo del suo ingente patrimonio. Lo stesso ordinario di diritto commerciale è indagato, perché, secondo il pubblico ministero, avrebbe manipolato un concorso ai danni di un ricercatore. Altre denunce penali sono attualmente in procura. Un'università che ha perso circa 200 posizioni nei *ranking* internazionali, come sottolineato anche dal «Corriere della sera». Passiamo al policlinico universitario: decine e decine di rimborsi per contenzioso, quasi 5 milioni di euro (lo ha detto «la Repubblica» pochi mesi fa). Una *performance* così bassa che è quattro volte peggio della media nazionale, non certo per colpa di chi ci lavora. Un'azienda con un *deficit* che ha toccato punte di 70 milioni di euro e che si è ridotto a 24 milioni di euro con tagli mostruosi. Si cade dalle barelle e si muore, solo la scorsa settimana; ma casi del genere sono avvenuti anche nel 2018, nel 2017 e ancora indietro. Fuga del personale: solamente nel reparto di cardiologia sono fuggiti dieci cardiologi. Non sono sorpreso, visto che il cardiologo in oggetto è lo stesso della puntata di «Report» ed è lo stesso che disse a me che ognuno ha il suo mandamento. Lo stesso policlinico è oggetto di varie interrogazioni (la faccio breve e concludo); tali interrogazioni, così come le denunce penali, avranno risposte, già date dalla giustizia amministrativa. Ma il punto non è questo. Il punto è che chi alza la testa viene minacciato: è successo al ricercatore autore della lettera ed è successo al sottoscritto, dichiarato "morto" dal direttore generale e dal rettore, il sottoscritto non avrebbe più trovato posto in nessuna parte d'Italia. Beh, non sono morto e sono resuscitato qui, in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lasciamo perdere il necrologio che mi è stato inviato nel 2017; lasciamo perdere le recenti minacce che hanno che hanno raggiunto mia moglie nelle settimane scorse (indirette, ma sempre minacce sono). Bene, in questo clima di paura e di omertà diffusa quando qualcuno alza la testa, esistono ricatti, vendette, intimidazioni ed emarginazione, *modus operandi* *modus operandi* tipico di una consorteria che uccide senza sparare. Ma lo Stato è vicino a coloro che alzano la testa e oggi ancor di più. Solo chi è parte di un sistema malato vuole difendere a tutti i costi quel sistema, praticando e continuando in pratiche poco chiare. Fatemelo dire e concludo: questo è un cancro e il cancro si elimina solo estirpandolo e curandolo. Se non lo curi, il cancro uccide il corpo intero, ma proprio per la sua irregolare, invasiva e anarchica natura, irrispettosa dei tessuti circostanti, uccide il corpo senza sapere che morirà insieme ad esso. Per rispetto dell'etica e di tutti, per rispetto del popolo italiano, invito rettore, prorettore e direttore generale a dimettersi per dare l'esempio all'Italia.

un terremoto che fece più di 300 morti, 70.000 sfollati e che a cinquantuno anni di distanza ancora non ha visto da parte dello Stato tutto l'intervento necessario per la ricostruzione. Stamattina il sindaco, il consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali del Comune di Santa Margherita del Belice hanno riunito un consiglio comunale straordinario in piazza Montecitorio per rassegnare la protesta civile di un popolo intero per la situazione in cui ancora si trova questa importante parte della Sicilia. Immaginate che in quel comune vi è ancora un quartiere di 200 famiglie dove non vi è l'acqua, non vi è l'energia elettrica, non vi sono le fognature e non vi sono le strade. Ritengo che una società civile debba interessarsi a una vicenda come questa, non dimenticando che, a fronte degli 8 miliardi di euro che sono stati spesi per la ricostruzione di tutto il Belice, lo Stato ha incassato in questi cinquantuno anni, con 27 provvedimenti legislativi, oltre 26 miliardi di euro di accise. Questi sono dati incontrovertibili

come impegno inderogabile di solidarietà, debba diventare patrimonio comune di quest'Assemblea. È un invito anche al Governo e alle forze parlamentari, perché si dia quanto prima una risposta a questi nostri fratelli siciliani. *(Applausi

un'intera amministrazione comunale, dal centrodestra fino al centrosinistra, maggioranza e opposizione, si è recata dinanzi a Montecitorio per lanciare un grido d'allarme scandaloso: anni ci sono ancora 200 famiglie che non hanno l'acqua, che viene portata loro con le botti, non hanno l'illuminazione e addirittura vi sono cento famiglie che ancora devono percepire i soldi per la ricostruzione delle loro case. Questi signori, nostri concittadini, si aspettavano dal Governo del cambiamento - non soltanto dal Governo e dalla maggioranza, ma dall'intero Parlamento - finalmente la parola «fine» al loro disagio nell'ultima legge di bilancio. Qui ci sono tanti esponenti di maggioranza eletti di quel territorio; mi rammarica il fatto che non vi sia stato nessun provvedimento che almeno denunciasse questa vicenda.

come ha detto bene chi mi ha preceduto, noi paghiamo tante tasse sulla benzina. Il Governo di Aldo Moro, negli anni Settanta, introdusse dieci lire sul costo di un litro di benzina.

Dove vanno tutti questi soldi? Questo è il quesito che noi dobbiamo porci. Non dobbiamo ingannare l'opinione pubblica mantenendo queste accise, perché sono francamente destituite di ogni fondamento, se non vanno

All'interno del tessuto urbano comunale sono presenti ben 12 stabilimenti industriali di categoria RIR (a rischio di incidente rilevante). Questo numero fa di Genova la seconda città del Paese per numero di attività industriali pericolose. In particolare, quattro di queste attività sono industrie petrolchimiche, che si trovano nel Ponente genovese, all'interno del quartiere di Moltedo, in cui abitano circa 5.000 persone; nel raggio di 5 chilometri da esse, si conta una popolazione di più di 100.000 abitanti. Questi stabilimenti movimentano sostanze chimiche e prodotti cancerogeni. In questi ultimi decenni sono stati numerosissimi gli esposti e le segnalazioni da parte della cittadinanza e dei comitati, per denunciare le criticità ambientali dovute all'inquinamento atmosferico o del suolo. Dopo una serie di incidenti, alla fine degli anni Ottanta si giunse a un protocollo d'intesa che avrebbe dovuto portare alla cessazione o al ricollocamento di alcuni di questi impianti entro il 1991. L'anno successivo, nel 1992, la Regione approvò un piano territoriale con i medesimi obiettivi. Identici obiettivi furono quelli del comitato tecnico regionale nella seduta del 2015. Oggi, nel 2019, e negli ultimi trent'anni, la politica locale ha derogato e disatteso le stesse regole che si era data. Anche il nuovo sindaco, Marco Bucci, volendo, a suo dire, distaccarsi da un precedente *modus operandi* politico, ha dichiarato qualche mese fa che avrebbe, entro poco tempo, preso una decisione in merito a questi stabilimenti e che, di conseguenza, avrebbe risolto l'annosa situazione. Personalmente spero che, dopo tutti questi anni, si possa finalmente tenere in conto le esigenze dei cittadini, che da anni si battono per il loro ambiente e il loro territorio. Sono certo che si debba arrivare, nel tempo che ci separa da una soluzione radicale di queste problematiche, a una capillare campagna di monitoraggio ambientale, che fino a oggi non è stata esercitata in maniera sufficiente, anzi, è stata assolutamente parziale e non continuativa nel tempo. La finalità dovrà essere quella di raccogliere, in maniera trasparente ed efficace, campioni e dati riguardanti la concentrazione di sostanze inquinanti nel territorio interessato. Da Roma saremo sicuramente attenti e faremo di tutto affinché gli enti locali garantiscano il diritto alla salute dei miei concittadini.

Signor Presidente, credo che in questi giorni siamo stati tutti contenti della cattura del terrorista comunista Cesare Battisti. Ma se tutto ciò è avvenuto, credo che lo si debba molto al cambio di Governo del Brasile e alle elezioni del nuovo presidente Bolsonaro. Ricordo che il precedente Presidente, come ultimo atto del suo mandato, aveva firmato per l'esatto contrario: per tenere ben saldo e soprattutto libero il terrorista.

Ci tengo anche a dire che mi aspetto da certi intellettuali o pseudointellettuali - da Vauro a Saviano - che chiedano scusa ai parenti delle vittime, perché, cari colleghi, per loro

Signor Presidente, prendo la parola per anticipare la presentazione di un'interrogazione da parte del mio Gruppo in relazione alle immagini apparse su alcuni quotidiani e televisioni, che mostravano il signor ministro della giustizia Bonafede indossare la divisa del corpo di Polizia penitenziaria, atteggiamento già peraltro più volte esibito in modo reiterato dal ministro dell'interno Salvini con la divisa della Polizia di Stato

che il Ministro stia indossando abusivamente e in pubblico segni distintivi di un corpo e di una professione senza averne titolo. Il Ministro non è abilitato ad indossare la divisa del corpo di Polizia penitenziaria, del quale non è un appartenente. Il Ministro ha responsabilità politiche, direttive, di governo, ma questo non lo abilita ad una professione, né tantomeno ad indossarne i simboli e la dotazione. Il Ministro viola la dignità delle istituzioni indossando fregi che non gli competono. Ripeto, il Ministro non è un appartenente al corpo di Polizia penitenziaria e la sua condotta, oltre a violare l'articolo 498 del codice penale, rischia di banalizzare la divisa come fosse un costume. La divisa è molto di più: è appartenenza; è servizio allo Stato e ai cittadini; è responsabilità di funzioni; è abnegazione nell'adempimento di compiti quotidiani. Ci sono modi concreti e meno propagandistici di dimostrare la vicinanza agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria, per esempio adoperandosi per migliorare le condizioni di lavoro, di funzionamento degli istituti penitenziari, aumentando le unità in servizio, aggiustando anche alcuni aspetti del riordino e riallineamento che avevamo avviato nella scorsa legislatura. Si occupi della grave carenza di approvvigionamento del vestiario, degli orari e delle condizioni di servizio, troppo spesso caratterizzati da violenze e aggressioni all'interno degli istituti, condizioni di stress che spesso portano al suicidio o a tentativi di suicidio degli appartenenti al Corpo. Si occupi il Ministro delle condizioni per la rieducazione della popolazione detenuta e per il reinserimento sociale dei condannati. Presidente, la sicurezza è un bene, è un diritto primario che non può essere strumentalizzato. Non siamo in un videogioco, siamo uomini e donne delle istituzioni: sobrietà, rispetto ed autorevolezza non possono essere svenduti al consenso, né ad esso essere

prendo la parola a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle per manifestare tutto il nostro disagio e disappunto per l'organizzazione di una mostra celebrativa

mancano tante foto e noi dobbiamo ricordarle. Per prime vanno ricordate quelle dei sodali di Andreotti: manca la foto di Salvo Lima, dei cugini Nino e Ignazio Salvo, ma mancano soprattutto le foto delle vittime della mafia. Manca la foto di Piersanti Mattarella.

che Cosa nostra si apprestava a compiere. Andreotti ha discusso con la cupola del delitto Mattarella prima che questo avvenisse e poi è tornato in Sicilia, dopo il delitto, per discuterne ancora e rimproverarli, perché non avevano fatto come diceva lui. Noi da questa storia prendiamo le distanze. Non ci troviamo nulla di celebrativo. È un'offesa per il nostro Paese, è una offesa alla memoria dei nostri morti e anche per il Presidente della Repubblica. Chiudiamo questa mostra subito! *(Applausi dal

che per noi l'arresto di Cesare Battisti chiude una ferita per tutti gli italiani, per la nostra Repubblica

tutti i Governi hanno profuso lo sforzo massimo per arrivare a questo risultato. Anche noi vogliamo ringraziare le Forze dell'ordine, in particolare la Polizia e il suo capo, per questo risultato così importante. Signor Presidente, in un'Italia che mai, in un'Italia che mai, soprattutto in un momento come questo, può subire la mistificazione della storia, sappiamo che il terrorismo di qualunque natura è stato sconfitto perché le forze democratiche e, soprattutto, i comunisti italiani,

suo nome un aggettivo: quando c'è di mezzo il terrorismo, qualunque connotazione rischia di essere sbagliata. Il terrorismo è criminale sempre. Lo abbiamo sconfitto perché lo abbiamo considerato senza alcuna ambiguità. Quando al nome di Cesare Battisti viene accostata la parola comunista, forse si fa un favore a Cesare Battisti, ma certamente si fa un torto a milioni di comunisti italiani che hanno combattuto strenuamente il terrorismo in Italia. Si fa un torto a tanti familiari delle vittime, alla memoria e all'impegno dell'operaio comunista Guido Rossa, trucidato dai terroristi nel nostro Paese.

e dai familiari colpiti dai crimini di Cesare Battisti; quell'esempio e quella dignità che, a mio avviso, non hanno nulla a che spartire con il circo mediatico imbastito nelle scorse ore, la cui sobrietà, il cui richiamo invece allo Stato di diritto niente ha a che spartire con chi cerca di strumentalizzare la vicenda per qualche voto; quello Stato di diritto che è l'esempio a cui tutti noi ci dobbiamo richiamare per dare la lezione più forte a chi, come Cesare Battisti, quello Stato, le nostre istituzioni e il nostro popolo ha voluto infangare. Non dobbiamo più permetterlo.

Non voglio però parlare di questo, ma del fatto che il senatore Giarrusso ha potuto esprimere liberamente la propria opinione, come lo posso fare io, grazie all'esistenza di Giulio Andreotti

Giarrusso, non riconoscere che cosa ha fatto Andreotti con Pecchioli, con Bachelet, nella lotta al terrorismo durante gli anni in cui ho vissuto direttamente quell'esperienza. Sono fatti Sono fatti storici e degli uomini hanno garantito a questo Paese di essere nel mondo occidentale, di avere le garanzie di libertà e ponendolo anche come riferimento dei Paesi del Medio Oriente. Non voglio dimenticare che cos'è la politica estera che ha posto l'Italia al centro dell'Europa: questo grazie alla politica estera di Andreotti e di Moro. Sono cose che ciascuno di voi e ciascuno di noi sa, e allora arrivare alla meschinità di dimenticare tutto questo per arrivare a un'azione politica di piccolo cabotaggio